il senatore Di Giovan Paolo ha chiesto informazioni e chiarimenti su un tema particolarmente delicato e che il Governo considera importante: la tratta degli esseri umani e la Convenzione di Varsavia del 16 maggio 2005. La Convenzione, com'è noto, è stata firmata dai Capi di Stato e di Governo di numerosi Paesi membri del Consiglio d'Europa durante il vertice di Varsavia del maggio del 2005. Tra l'altro, nella fase del negoziato, sappiamo che l'Italia è stata tra i maggiori sostenitori e propulsori della Convenzione, nella consapevolezza di quanto fondamentale sia una disciplina uniforme del fenomeno della tratta in ambito europeo, perché non vi siano zone franche rispetto a questo fenomeno abominevole già regolato e punito severamente nel nostro ordinamento. infatti, rilevare che la nostra Nazione, avendo già ratificato con la legge n. 146 del 2006 il Protocollo di Palermo e l'annessa Convenzione ONU sul crimine transnazionale organizzato, ha già recepito nel proprio ordinamento la definizione di tratta accolta nella Convenzione di Varsavia, come pure ha già messo in atto l'impegno a punire le condotte criminose connesse alla tratta così definita con sanzioni adeguate, proporzionate ed efficaci. La legge n. 228 del 2003 recante misure contro la tratta di persone, modificando le disposizioni degli articoli 600 e 601 del codice penale, ha poi recepito le prescrizioni contenute nel Protocollo di Palermo, ricollocando le condotte criminose da questo ultimo previste all'interno dei delitti contro la schiavitù. In particolare, ricordo che l'articolo 600 del codice penale punisce con la reclusione da otto a venti anni chiunque riduce o mantiene in schiavitù una persona costringendola a prestazioni lavorative sessuali o a prestazione che ne comportino lo sfruttamento, mentre l'articolo 601 del codice penale punisce con la reclusione da otto a venti anni chiunque costringa una persona a fare ingresso, soggiornare o ad uscire dal territorio dello Stato riducendola in condizione di schiavitù. Ugualmente deve dirsi per le disposizioni della Convenzione inerenti le misure investigative e processuali per contrastare il fenomeno della tratta, per le quali la legge n. 228 del 2003 e la successiva legge n. 146 del 2006 hanno già predisposto strumenti adeguati, tali da considerare rispettati gli standard imposti dal Consiglio d'Europa. Quanto alle misure di protezione, assistenza e sostegno previste a favore delle vittime di tratta, il nostro sistema normativo, costituito dall'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione e dalla legge n. 228 del 2003 e relative norme di attuazione, consente che alle persone vittime di tratta siano fornite misure di sostegno e protezione, sia nell'ambito di programmi di cosiddetta prima accoglienza (i programmi *ex* articolo 13 della legge n.

e persegue entrambi gli obiettivi in esse indicati: rafforzare la repressione del traffico di persone e tutelare le vittime. La protezione delle vittime diviene dunque momento qualificante, non soltanto non incompatibile con il contrasto delle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di persone per finalità di sfruttamento, ma addirittura sinergico rispetto all'attività repressiva. Le vittime di tratta possono accedere ai programmi di assistenza ed è loro rilasciato, come tutti sapete, un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi, rinnovabile per un ulteriore anno. Sulla base di queste considerazioni, riteniamo quindi che il nostro ordinamento sia già in linea con gran parte delle disposizioni contenute nella Convenzione di Varsavia. Anche l'ultimo rapporto degli Stati Uniti sulla tratta (una ricerca che ha incluso 149 Paesi), si è espresso in modo favorevole nei confronti dell'Italia, inserendola tra i Paesi virtuosi e apprezzando, in particolar modo, la norma contenuta nel più volte citato articolo 18. Allo scopo, comunque, di verificare la necessità di procedere ad ulteriori interventi normativi in ordine ad un tema che, come ho detto prima, il Governo considera estremamente delicato e rilevante, il Ministero degli esteri ha avviato i necessari contatti con le amministrazioni interessate, tra cui il Ministero per le pari opportunità, impegnato in prima linea contro la tratta, al fine di costituire un tavolo di lavoro finalizzato ad individuare eventuali princìpi, contenuti nella Convenzione di Varsavia che ancora necessitino di recepimento. Peraltro, non manca un impegno costante del Ministero per le pari opportunità, sia per il recupero delle vittime di tratta, al fine di sostenerle in un percorso di reinserimento nella vita sociale, sia nel contrasto delle organizzazioni criminali che riducono in schiavitù le proprie vittime. Tra le misure intraprese all'inizio del mio impegno governativo, ho provveduto a ricostituire la Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento, e cioè l'organo che svolge la funzione di sovrintendere all'erogazione ed al controllo dei finanziamenti statali per la realizzazione dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime. La Commissione, in primo luogo, ha provveduto, il 5 agosto 2008, ad adottare il bando pubblico per l'erogazione dei finanziamenti statali, nella misura di 2,5 milioni di euro, destinati ai programmi di prima assistenza a favore delle vittime dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale (quindi vittime dei reati di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani), finalizzati a garantire, in via transitoria, alle vittime dei reati anzidetti adeguate condizioni di alloggio, vitto ed assistenza sanitaria. In secondo luogo, la Commissione interministeriale ha provveduto a definire il contenuto di un ulteriore bando, pubblicato nel febbraio 2009, per il finanziamento dei programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione, finalizzati a dare alle vittime della tratta l'opportunità di affrancarsi dai circuiti di sfruttamento ed iniziare un percorso per il recupero di condizioni normali di vita e l'integrazione nel tessuto sociale italiano. Ricordo inoltre che, soprattutto pensando alla condizione delle persone vittime di tratta, costrette a vivere nella clandestinità e in una condizione di maggiore dipendenza, sia psicologica che fisica dai propri trafficanti, ho voluto introdurre nel disegno di legge recante misure contro la prostituzione, in discussione al Senato, la nuova fattispecie criminosa dell'associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. Quasi sempre, infatti, dietro alla prostituzione si nasconde un'organizzazione criminale che riduce in schiavitù le proprie vittime: il reato di sfruttamento della prostituzione, di riduzione in schiavitù o di tratta di esseri umani deve essere affiancato da una specifica previsione di associazione per delinquere, quando questa è diretta allo sfruttamento della prostituzione. Per contrastare le organizzazioni finalizzate al compimento di reati di sfruttamento della prostituzione minorile e di induzione e favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione, è previsto nel disegno di legge un inasprimento delle pene per questo tipo di associazione a delinquere, stabilite nella reclusione da quattro a otto anni per i promotori e gli organizzatori dell'associazione, e da due a sei anni per i partecipanti. Le informazioni fin qui fornite confermano l'impegno e l'attenzione del Ministero per le pari opportunità sul fenomeno della tratta degli esseri umani, impegno che peraltro è di tutto il Governo. Non si può e non si deve abbassare la guardia su un tema così rilevante, ma occorre continuare a spiegare sempre maggiori energie per combattere un fenomeno strettamente collegato a quello dell'immigrazione clandestina, come dimostrano anche i recenti dati forniti dalla Croce Rossa italiana sull'ingresso di vittime minorenni ridotte in condizioni di piccoli schiavi. Ho detto che non si può e non si deve abbassare la guardia: non lo abbiamo fatto, non lo stiamo facendo e non lo faremo. Vi ringrazio per l'attenzione.

Credo che, date le condizioni, questo sia l'ambiente più sereno per mostrare che siamo avversari politici, non nemici, signora Ministro, nel senso che abbiamo un'idea diametralmente opposta alla vostra rispetto a questo e le spiegherò perché, con grande rispetto per lo sforzo che compie; anzi, le dico sin d'ora che saremo al suo fianco, considerando che tutte le sue iniziative - che sono lodevoli e che condividiamo - sono sostanzialmente azzerate dai tagli

perché ritenete che sulla tortura si sia già in una fase di copertura. Per carità, è legittimo, perché il dibattito su questo punto è aperto, però bisogna dire con molta chiarezza che

cioè a colui che ha battuto il presidente Berlusconi due volte, formando due Governi nei quali le scelte dell'articolo 18 della legge n. 228 del 2003 a protezione della vittima

con la sua collega Prestigiacomo) hanno ritenuto di attuare una legge che era condivisa rispetto a questo problema. Allora, il primo dato è questo: se non intendete ratificare le Convenzioni, non c'è nessuno scandalo, però ditelo con chiarezza, perché ritenete che siamo già in copertura, dal punto di vista delle norme. In secondo luogo, un rischio forte c'è: ho partecipato alla seduta in cui lei ha presentato il programma del suo Ministero nella Commissione affari costituzionali di questo ramo del Parlamento. di un programma assolutamente condivisibile, purtroppo però falcidiato - come dicevo prima - dall'assenza di attenzione dal punto di vista economico, con il rischio che venga massimizzata la retorica rispetto alla difesa dei soggetti deboli e minimizzata la portata delle Convenzioni e delle azioni positive in questo campo.

in nulla, ha sempre inteso assumere scelte liberali in questi campi, non esercitare una compassione che non ha nulla a che fare con la politica. La politica è messa in sicurezza dei deboli attraverso l'esercizio dei diritti riconosciuti e non attraverso l'esercizio della carità e della compassione nei confronti dei più deboli. Sono due cose diverse: una è la testimonianza, l'altra è la politica. Concludo l'immigrazione, la prostituzione, le questioni legate ai minori sono strettamente connesse alla tratta degli esseri umani, che è la moderna schiavitù. Su questo siamo d'accordo, ma se noi non rinforziamo la dotazione economica a disposizione dei poteri locali, la dotazione economica a disposizione delle associazioni che sul campo, nella società civile, nei corpi intermedi (non solamente lo Stato nella sua più alta espressione o i Ministeri) operano tutti i giorni, diamo una risposta semplicemente retorica. Ora, ci sarà modo e possibilità di ritornare sul tema della prostituzione. Lo faremo e ci confronteremo, ma con molta tranquillità. Io volevo dirle che la nostra è un'idea diversa, perché noi riteniamo che le Convenzioni vadano ratificate, soprattutto quando sono state firmate. Il nostro Paese le ha firmate e dovrebbe ratificarle.

per i beni e le attività culturali*. Signora Presidente, con riferimento al problema rappresentato dall'interrogante, senatore Marcucci, si riferisce quanto segue. L'intervento di restauro e riallestimento del Museo garibaldino di Caprera è stato inserito nella programmazione triennale dei Fondi Lotto

La rimodulazione operata dal Ministero per i beni e le attività culturali, a seguito delle modifiche di bilancio introdotte sia dalla legge finanziaria n. 244, sia dalla recente manovra finanziaria, non ha intaccato lo stanziamento per il 2007 (che ricordo essere pari essere pari a 537.000 euro) ed ha, invece, previsto la revoca delle risorse del 2008 sulla programmazione Lotto ed il contestuale rifinanziamento a valere sulle risorse previste

Per il 2009 è stato, invece, assicurato uno stanziamento di 194.650,86 euro sempre sul programma Lotto. Relativamente alla questione posta dal senatore Marcucci circa la revoca dell'intera somma destinata per il 2008, pari a 553.420 euro, si specifica che, essendo stato l'intervento contestualmente rifinanziato con altre risorse, il finanziamento per il 2008 non è stato revocato ma ridotto di 117.891,80 euro, passando quindi dagli iniziali e previsti 553.420 euro

Si fa infine presente che, alla luce della rimodulazione effettuata, le risorse complessivamente assegnate al Compendio garibaldino di Caprera sono pari a 1.167.000 euro, a fronte dei previsti 1.649.000 euro.

*(PD)*. Signora Presidente, signor Sottosegretario, credo si debba partire dal 2007, l'anno del bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi. A quell'epoca, il Governo Prodi, con sensibilità, decise d'intervenire sul Compendio garibaldino di Caprera (che, lo ricordo, è il vero sacrario laico dell'Unità d'Italia) proprio perché nel tempo tale

con riferimento all'interrogazione del senatore Vita, si rappresenta quanto segue. Le linee strategiche di azione del Ministero per i beni e le attività culturali sono prioritariamente indirizzate verso una gestione dinamica del patrimonio e delle attività culturali che, ferma restando la priorità della tutela, sappia valorizzare al meglio le enormi potenzialità in essi contenute e, forse, non adeguatamente espresse, anche al fine di sviluppare sinergie con altri settori produttivi del Paese. In tale ambito sono già state poste in atto alcune profìcue iniziative di collaborazione tra il settore pubblico e quello privato per l'attuazione di nuovi modelli di gestione e di valorizzazione del ricco patrimonio culturale ed artistico italiano, sia in attuazione delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, sia secondo metodologie sperimentate con successo in altri Paesi. Per perseguire con maggiore incisività, efficienza ed efficacia questa linea d'indirizzo e di azione è stata individuata in particolare, quale precipua priorità politica del Ministero, la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale italiano, anche all'estero. Lo sviluppo di tale settore è volto, da un lato, a garantire quale servizio ai cittadini, una maggiore conoscibilità e fruibilità dei beni e, dall'altro ad attrarre, quale strumento di sviluppo economico, investimenti da parte dell'imprenditoria culturale. A tal fine, si è ritenuto necessario avvalersi dell'apporto professionale del dottor Mario Resca, il quale è stato nominato consigliere del Ministro per la valorizzazione dei musei, con decreto in data 25 novembre 2008, registrato dal competente organo di controllo in data 10 dicembre 2008, al numero 847. Il predetto incarico è a titolo gratuito. Sempre nell'ottica di accrescere e di sviluppare coerentemente su tutto il territorio nazionale le potenzialità, anche economiche, del sistema museale nazionale, lo schema di regolamento di modifica al decreto del del 2007, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 18 dicembre 2008 ed attualmente all'esame del Consiglio di Stato, prevede, fra l'altro, l'istituzione, all'articolo 8, della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. A tale Direzione sono attribuite competenze trasversali in materia di promozione della conoscenza, fruizione pubblica e valorizzazione del patrimonio culturale, ed ai luoghi della cultura di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato, ferme restando le competenze in materia di tutela e salvaguardia del patrimonio stesso attribuite in via monocratica ed esclusiva, *ex* articolo 9 della Costituzione, alle strutture che svolgono funzioni di carattere tecnico-scientifico. In tale contesto, l'esperienza e la professionalità altamente qualificate e le specifiche capacità manageriali del dottor Resca rappresentano un indubbio valore aggiunto per il raggiungimento degli obiettivi illustrati, che il Ministero per i beni e le attività culturali intende perseguire nel settore, in stretta collaborazione con le eccellenti professionalità tecniche e scientifiche da sempre presenti nel Dicastero attraverso le Sovrintendenze statali, che costituiscono la più illustre tradizione in materia di attività di tutela e di restauro del patrimonio culturale, riconosciuta ed apprezzata in tutto il mondo.

per aver illustrato una risposta che certo è il frutto di una riflessione degli uffici del Ministero. Aggiungo, senza nulla dire delle persone (in questo caso di Mario Resca), che ciò che spinse alcuni di noi, tra cui il collega Marcucci che siede accanto a me, a presentare, a suo tempo, questa interrogazione fu il vasto moto di protesta che emergeva dall'insieme degli operatori, dei professionisti, degli intellettuali ed anche dei direttori, dei funzionari e degli addetti dello stesso Ministero. Infatti, l'avvento del dottor Resca costituiva

indagare semanticamente sul punto di contatto o sul punto di asimmetria tra tutela e valorizzazione (scopriremmo dopo qualche ora di intenso seminario che i due concetti stanno assieme), ma, proprio per questo, aver immaginato una direzione figlia un po' della cultura mercatista e liberista di un'altra fase del mondo, quella che, com'è noto, precedette lo sconquasso attuale, è sembrato è sembrato non tanto e solo agli interroganti, ma a tanta parte della cultura italiana una rottura, non della continuità (la continuità può essere interrotta) ma di una tradizione, quella migliore, che ha animato il nostro Paese nella difesa e nello sviluppo del suo immenso patrimonio culturale; tant'è vero che la reazione è stata piuttosto consistente e il dibattito pubblico assai aspro. Per concludere, vorrei fare una considerazione di merito. Sono passati ormai dei mesi,

sloganistica nell'attività culturale quasi a far sperare, intuire o temere (a seconda dei punti di vista) che ci fosse un'improvvisa apertura al mercato e del mercato,

una visione un po' leggera e troppo modaiola dei termini e delle scelte che riguardano un intero apparato della vita pubblica italiana; per un altro, non rispondere invece al capitolo essenziale delle risorse che mancano

Signor Presidente, l'onorevole senatore interrogante fa presente che per l'inquadramento nel profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi l'amministrazione ha applicato norme di ricostruzione di carriera diverse a seconda che l'inquadramento in tale profilo sia avvenuto prima o dopo il 2003 ed ha così determinato un trattamento disomogeneo.

è stato definito il profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi. Con lo stesso articolo è stato altresì previsto,

Le modalità di ricostruzione della carriera e di collocazione nel profilo sono state definite a mezzo dei contratti nazionali del comparto scuola del 2001 e del 2003. Per effetto dell'articolo 8 del contratto del 2001 al personale in questione è stato riconosciuto, con decorrenza dal 1° settembre 2000, in aggiunta allo stipendio iniziale del profilo di provenienza, un incremento retributivo pari al 70 per cento del differenziale tra la posizione stipendiale del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo. È stata altresì prevista, dal comma 2 dello stesso articolo, l'assegnazione di una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell'eventuale assegno *ad personam* nonché del rateo di anzianità in corso di maturazione e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. Sulla base degli incrementi stipendiali succitati, gli stessi DSGA sono stati inquadrati nel profilo professionale con il criterio della temporizzazione, così come previsto dal successivo comma 3, del suindicato articolo 8 del CCNL del 2001. Con il successivo contratto del 24 luglio 2003 è stato attribuito un ulteriore 30 per cento del succitato differenziale ed è stata quindi conseguita la totale equiparazione retributiva tra gli ex responsabili amministrativi ed i direttori di accademia e di conservatori. A seguito di tale equiparazione sono state nuovamente definite le posizioni stipendiali, utilizzando sempre il medesimo criterio della cosiddetta temporizzazione. Il personale in questione chiede che l'inquadramento nell'area contrattuale "D" sia nuovamente effettuato in applicazione delle modalità previste dall'articolo 66, comma 6, del CCNL 1995 che prescrive, per la ricostruzione della carriera, il riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo. Il periodo prestato in qualità di responsabile amministrativo, ad avviso degli interessati, deve essere considerato come servizio prestato in ruolo diverso rispetto a quello della nomina a DSGA. I predetti invocano, in sostanza, il pieno riconoscimento giuridico ed economico, alla data del 1° settembre 2000, dell'anzianità maturata al 31 agosto 2000. L'amministrazione non ha accolto le richieste di inquadramento difformi rispetto alle norme citate anche perché a seguito dell'entrata in vigore dell'autonomia scolastica, di cui alla legge n. 59 del 15 marzo 1997, il profilo di responsabile amministrativo, come innanzi evidenziato, è stato abolito e trasformato in quello di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Tale figura è apicale, così come lo era quella del responsabile amministrativo, tanto è vero che non è stata prevista l'effettuazione di alcun periodo di prova all'atto dell'inquadramento nella nuova qualifica, mentre il riconoscimento del servizio di ruolo prestato nella carriera inferiore, ai sensi dell'articolo 66 del CCNL del 1995, è attribuito agli assistenti amministrativi, nominati nella qualifica di DSGA a seguito del superamento di concorsi selettivi banditi specificatamente e che, appunto, devono superare il periodo di prova. In proposito anche l'ARAN, a fronte della richiesta di questo Ministero per l'eventuale "interpretazione autentica" delle norme contrattuali in questione, con nota del 21 aprile 2005, ha ribadito che il passaggio di profilo del personale in questione non può configurarsi come passaggio tra ruoli differenti bensì come '"...trasformazione, senza soluzione di continuità, dal profilo professionale di Responsabile amministrativo a direttore dei servizi generali e amministrativi...", escludendo, quindi, la possibilità del pieno riconoscimento giuridico ed economico, alla data dei 1° settembre 2000 (decorrenza nomina DSGA), dell'anzianità maturata al 31 agosto 2000 in qualità di responsabile amministrativo. A decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 l'amministrazione, per l'inquadramento in ruolo dei nuovi DSGA, ha previsto, secondo regola, il riconoscimento del servizio prestato dai medesimi in qualità, appunto, di assistenti amministrativi. In tale nuova situazione i medesimi pongono eccezione di disparità di trattamento. In proposito va ribadito che le disposizioni relative alla gestione del passaggio dei responsabili amministrativi alla figura di direttore dei servizi generali e amministrativi si pongono come *lex specialis* che, in quanto tale, risulta, per sua natura, esclusiva di qualsiasi altra norma concorrente di carattere generale, quali sono, appunto, le norme generali sulle ricostruzioni di carriera. Va inoltre considerato che tale disciplina appare, ancor più, come norma speciale in quanto inserita nel contesto di contratti collettivi nazionali di comparto e cioè di strumenti normativi di valenza tecnico-giuridica che non solo assurgono a pieno titolo al rango di fonte primaria, ma che inoltre trovano fondamento ed efficacia nella sintesi dell'accordo contrattuale stipulato tra la parte pubblica e la parte sociale. Infine, in merito alla richiesta dell'onorevole senatore interrogante su quali siano i provvedimenti che il Ministero intende adottare, va precisato che, al fine della eventuale revisione dell'inquadramento già disposto, si è provveduto a quantificare l'onere aggiuntivo con effetto *ex nunc*, poiché la revisione in oggetto non dovrebbe comportare la corresponsione di alcun arretrato. Questa valutazione è stata assunta con l'evidente proposito di riesaminare la questione, compatibilmente con le esigenze di bilancio, in sede di comitato di settore, in vista del prossimo rinnovo contrattuale del comparto scuola. Signora Presidente, ringrazio il Sottosegretario per questa risposta complessa

si risponde sulla base degli elementi riferiti dal rettore dell'Università della Basilicata e delle indicazioni fornite dalla competente direzione generale in merito alla gestione dell'ateneo nel rispetto delle normative vigenti. L'articolo 51, comma 4, della legge finanziaria per il 2008 stabiliva che le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non potessero eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul Fondo per il finanziamento ordinario. A determinare l'esatta individuazione delle partite di spesa fissa che concorressero a formare detto limite del 90 per cento era già intervenuto l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la quale disponeva che «in attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, per l'anno 2004, ai fini della valutazione del limite previsto dal suddetto articolo 51, non si tiene conto... dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università, previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002». Tale previsione, che introduceva un correttivo per detto limite e per l'anno 2004, veniva sostanzialmente confermata per i successivi esercizi finanziari fino al 2008 e, da ultimo, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10

Basilicata, a seguito delle verifiche disposte, anche per l'anno 2007, sulla base di quanto effettivamente speso per assegni fissi al personale di ruolo e di quanto considerato a valere sull'FFO, per effetto dei correttivi disposti annualmente per gli incrementi stipendiali annuali al personale di ruolo e ad altri costi per le procedure di stabilizzazione, risultava essere un ateneo virtuoso ed in perfetta linea con la normativa in vigore, avendo un rapporto certificato spese fisse-FFO pari all'87,84

individuava lo strumento di un piano programmatico, da approvarsi con provvedimenti interministeriali, per l'assegnazione di ulteriori risorse a valere sul Fondo di finanziamento ordinario. richiama disposizioni che rendevano effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni, ma nel solo caso degli atenei che avessero superato il predetto limite del 90 disposizione, peraltro, superata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito nella legge n. 1 del 2009. Fattispecie, questa, non riferibile all'Università della Basilicata, alla quale si applica, invece, la specifica disposizione di cui alla lettera c*-bis)* del suddetto comma 429. Si precisa che i finanziamenti erogati dalla Regione Basilicata all'ateneo lucano,

i finanziamenti regionali stanziati in favore dell'ateneo lucano costituiscono incrementi virtuali del Fondo di finanziamento ordinario derivanti da convenzioni stabili per la retribuzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi del già ricordato articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con legge 4 giugno 2004, n. 143, come specificato nella nota ministeriale, protocollo n. 686 del 21 aprile 2008. il Ministero, con nota del 17 novembre 2008, n. 1680, ha fatto presente che "i trasferimenti disposti dalla Regione Basilicata a favore dell'Università saranno considerati in aggiunta al Fondo di finanziamento ordinario in analogia a quanto già operato per tutti gli interventi di finanziamento stabile finalizzato all'assunzione di personale. Pertanto, i maggiori oneri derivanti dalla correlata programmazione non incideranno nel calcolo del limite del 90 per cento del rapporto tra assegni fissi e Fondo di finanziamento ordinario". La citata, ultima nota ministeriale ad oggetto la programmazione triennale degli oneri di personale per gli anni 2008-2010, nell'ambito della rilevazione, valida a livello nazionale, prevista dalla procedura PROPER-CINECA. Anche i competenti organi della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero dell'economia hanno confermato, per le vie brevi, tali circostanze. Il Rettore, da parte sua, ha anche riferito in merito alla popolazione studentesca dell'Università: ad oggi, gli immatricolati per l'anno accademico 2008-2009 risultano 2.165; l'andamento delle immatricolazioni presenta un sensibile e costante incremento proprio a partire dal 2006-2007, risultando così in controtendenza virtuosa rispetto al *trend* nazionale che, sin dal 2002-2003, registra una costante flessione delle immatricolazioni stesse. Inoltre, il rapporto studenti-docenti è di 47 ad 1, se si considerano i soli professori in servizio, e diventa 28 a 1, ove si considerino anche docenti e ricercatori.

vale a dire la necessità che le università, in questo caso l'Università della Basilicata, non manchino di tener presente un equilibrio virtuoso tra le risorse

un'azione sproporzionata di allargamento dell'organico, sottraendo invece utili risorse a progetti di ricerca che aumentino anche la qualità della stessa Università

gestiti dalla società "Istituto Studium s.r.l", affermando che la vicenda stessa si sarebbe determinata per la "mancanza di un sistema adeguato di controllo e valutazione delle scuole private paritarie". Per quel che riguarda la vigilanza, le vigenti norme in materia di parità scolastica - la legge n. 62 del 2000, l'articolo 1-*bis* della legge n. 27 del 2006 regolamento adottato con il decreto ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007, recante la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento prevedono un'attività di vigilanza e controllo da parte degli uffici scolastici regionali sulla sussistenza e sulla permanenza dei requisiti richiesti per la parità scolastica. In particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto ministeriale, prevede che entro il 30 settembre di ogni anno i gestori delle scuole paritarie trasmettano all'ufficio scolastico regionale una dichiarazione attestante la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, nonché la documentazione relativa al funzionamento per l'anno scolastico in corso. Inoltre, il comma 4 dello stesso articolo dispone che "il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare e documentare tempestivamente all'ufficio scolastico regionale ogni eventuale variazione riguardante la gestione, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa ai fini delle conseguenti verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti prescritti." Per quel che riguarda poi la valutazione, ricordo che il decreto legislativo n. il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione ed ha affidato all'INVALSI specifici compiti in proposito, relativamente al sistema dell'istruzione, secondo gli indirizzi contenuti in apposita direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine, in questa legislatura, sono state emanate le direttive ministeriali nn. 74 e 75, entrambe in data 15 settembre 2008, riguardanti, la prima, la programmazione dell'attività dell'INVALSI per i tre anni scolastici decorrenti dal 1° settembre 2008, la seconda, gli obiettivi generali delle politiche educative nazionali per il corrente anno scolastico 2008/2009. Gli indirizzi contenuti nelle citate direttive si riferiscono indistintamente a tutte le scuole del sistema nazionale che, come è noto, è costituito dalle scuole paritarie private e degli enti locali, oltre che dalle scuole statali. Ciò preliminarmente precisato, vengo alla specifica vicenda descritta nell'interrogazione, relativa all'Istituto superiore paritario «Studium» di Milano. A tal proposito, la Direzione generale dell'ufficio scolastico della Lombardia ha trasmesso il decreto in data 8 settembre 2008, relativo alla revoca del riconoscimento della parità del ginnasio liceo classico «P. A. Gemelli» e del liceo scientifico «G. Marconi» di Milano. In questo decreto viene riportato che il 3 settembre 2008 «inopinatamente genitori di alunni dei suddetti licei ed organi di informazione denunciavano la mancata riapertura all'inizio dell'anno scolastico corrente dei medesimi licei» e che il 4 settembre il coordinatore didattico e l'amministratore unico della società "Istituto Studium s.r.l." «dichiaravano di non avere più la disponibilità dei locali e che l'acquisizione di una nuova sede non appariva immediatamente realizzabile». Nel medesimo decreto, comunque, veniva precisato che l'ufficio scolastico regionale avrebbe fornito assistenza alle famiglie affinché gli alunni potessero iscriversi a loro scelta presso istituzioni scolastiche statali o paritarie di Milano o Provincia dello stesso ordine e grado. In effetti, l'ufficio scolastico provinciale di Milano, con circolare dell'8 settembre 2008, ha disposto la riapertura delle iscrizioni per l'anno scolastico 2008/2009, in via del tutto eccezionale, esclusivamente per gli alunni provenienti dagli istituti in questione, autorizzando anche iscrizioni presso altre tipologie di indirizzo scolastico limitatamente agli alunni iscritti nelle prime classi. Il Ministero, da parte sua, per accertare lo svolgimento dei fatti e acquisire una dettagliata e circostanziata relazione sulla vicenda, ha disposto una indagine ispettiva che ha confermato quanto sopra e non ha rilevato inadempienze degli uffici della Direzione generale dell'ufficio scolastico regionale. Per quanto concerne il sistema di controllo e vigilanza nelle scuole della Lombardia, dalla relazione ispettiva risulta che, pur in presenza di un limitato contingente numerico di ispettori, sono state non di meno effettuate ispezioni su un significativo numero di istituzioni scolastiche della stessa Regione. In particolare, nelle scuole gestite dalla società «Studium», sono state effettuate quattro visite ispettive nell'arco di quattro anni e nell'anno scolastico 2006/2007 l'ispezione è stata effettuata dalla stessa coordinatrice degli ispettori della Lombardia. Quanto, infine, alle rilevate esigenze di personale ispettivo in Lombardia, tali esigenze saranno tenute ben presenti, comparativamente con quelle delle altre Regioni, in sede di assegnazione dei vincitori del concorso pubblico a 145 posti di dirigente tecnico,

in riferimento all'atto di sindacato ispettivo presentato dal senatore Ranucci e da altri senatori, si fa presente quanto segue. Gli eventi meteorologici che si sono verificati nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre sull'isola di Ventotene sono stati puntualmente monitorati dalla Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il Centro funzionale centrale, le Sale operative regionali, l'Ufficio territoriale di Governo e le strutture operative territoriali competenti. Inoltre si evidenzia che, a seguito dell'ondata di maltempo che ha interessato l'intera Penisola nei mesi di novembre e dicembre 2008, determinando fenomeni di dissesto idraulico, idrico ed ambientale, con conseguenti danni a strutture pubbliche e private e, in generale, una grave situazione dì pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, con decreto del Presidente del Consiglio del 18 dicembre 2008, è stata deliberata la dichiarazione dello stato di emergenza per tali eccezionali eventi meteorologici su tutto il territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2009. La successiva ordinanza di protezione civile n. 3734 del 16 gennaio 2009 ha provveduto a nominare commissari delegati per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi calamitosi, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ad essi è stato demandato il compito, previa individuazione delle Province e dei Comuni danneggiati, di accertare i danni, di adottare tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, di assicurare l'assistenza alle popolazioni colpite, nonché di porre in essere ogni utile attività per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione. In particolare, la suddetta ordinanza ha previsto che ciascun commissario delegato, relativamente al proprio ambito regionale, predisponga - sentiti i Comuni e le Province interessati - un piano generale degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità, comprensivo della quantificazione degli oneri. Nel piano sono compresi interventi per il ripristino della viabilità, delle infrastrutture, delle opere e dei servizi pubblici danneggiati, nonché per la pulizia, la bonifica e la manutenzione straordinaria degli alvei e delle opere di difesa idraulica dei corsi d'acqua interessati dagli eventi di piena. detto piano si prevede, inoltre, il ripristino delle funzionalità delle opere marittime di difesa della costa, la bonifica e la stabilizzazione dei versanti interessati da eventi franosi o valanghivi, nonché la realizzazione di ulteriori azioni ed opere di prevenzione e di mitigazione dei rischi ancora presenti o determinatisi a seguito degli avversi eventi meteorologici. È stato altresì disposto che ciascun commissario delegato ponga in essere ogni azione utile alla predisposizione, da parte dei Comuni esposti ad alto rischio idrogeologico ed idraulico, entro il termine di cessazione dello stato di emergenza, della pianificazione di emergenza, coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia. In riferimento, poi, ai provvedimenti relativi alle situazioni di rischio segnalate dall'onorevole senatore si fa presente che questi risultano inseriti nel piano di interventi predisposto dal commissario delegato della medesima Regione, ai sensi della suddetta ordinanza n. 3734. Infine, per quanto riguarda le misure a sostegno dell'economia del territorio dell'isola di Ventotene, si fa presente che la predetta ordinanza di Protezione civile ha previsto l'erogazione di una serie di contributi per favorire l'immediata ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate e, in particolare, un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature, comunque non superiore al 50 per cento del danno medesimo e fino ad un massimo di 200.000 euro; un contributo fino al 30 per cento del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e noi più utilizzabili, fino ad un massimo di 60.000 euro; nonché un contributo correlato alla durata della sospensione dell'attività, che non può eccedere i novanta giorni, quantificato in trecentosessantacinquesimi, sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata. In relazione alla situazione dei dissesti idrogeologici presenti sull'isola di Ventotene, si precisa che questa è stata inserita nel progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico adottato dalla Regione Lazio. In particolare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha destinato al Comune di Ventotene un finanziamento pari a 1,79 milioni di euro per gli interventi di consolidamento e messa in sicurezza della parete rocciosa del Porto romano. Gli interventi sono ad oggi in fase di progettazione.

è l'isola di Altiero Spinelli, dove egli ha avuto la straordinaria intuizione dell'Europa; è l'isola che ha delle aree marine protette molto importanti; è l'isola dove c'è

fatti sia per l'assetto idreogeologico sia per il ripristino delle strade. Ricordo che, ancora al 24 marzo 2009 - quindi, praticamente ieri - il sindaco di Ventotene è stato costretto emanare un'ordinanza in cui chiedeva la chiusura parziale, mediante opportuno transennamento del muro stradale, di via Cala Rossa per una lunghezza di 41 metri, il monitoraggio delle lesioni presenti sul muro

Signora Presidente, in riferimento all'atto di sindacato ispettivo presentato dalla senatrice Germontani, si fa presente quanto segue. Il giorno 7 giugno 2008 un violento nubifragio ha colpito la provincia di Parma, in particolare il comune di Varano de' Melegari, causando danni alle infrastrutture, alle abitazioni e l'esondazione del rio Raboni. Successivamente, con una nota del 25 giugno 2008, l'Amministrazione comunale di Varano de' Melegari ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile la richiesta d'intervento, approvata dal Consiglio comunale il 17 giugno 2008, trasmessa alla Regione Emilia Romagna ed agli altri enti istituzionalmente competenti, per il ristoro dei danni provocati dai predetti eventi meteorologici. Dall'analisi dei dati idropluviometrici, registrati presso il Centro funzionale centrale, non è stato, però, rilevato alcun valore significativo di precipitazione, né sono stati segnalati fenomeni di intumescenza dei corsi d'acqua ivi presenti. Inoltre non sono state riportate, sui mattinali della Sala situazioni Italia, notizie al riguardo. In particolare, si precisa che la Regione Emilia Romagna, con una nota del 24 giugno 2008, ha chiesto il riconoscimento dello stato di emergenza per eventi meteorici intensi verificatisi tra il 18 maggio ed il 15 giugno 2008 sul proprio territorio, non segnalando, tra questi, alcuna situazione di criticità nel periodo e nell'area oggetto della presente interrogazione. Allo stato degli atti, quindi, si ritiene che l'evento meteorologico segnalato abbia rivestito carattere di intensità solo a livello locale, con effetti al suolo ascrivibili ad uno scenario di criticità ordinaria e, pertanto, esso non può essere riferito ad eventi dì cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativo a «calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari». Per quanto riguarda i dissesti idrogeologici che si generano in conseguenza degli eventi meteorologici di elevata intensità, questi sono riconducibili a situazioni note da tempo e gli interventi necessari per loro soluzione risultano in gran parte già pianificati. Purtroppo, l'esiguità delle risorse disponibili non ha finora permesso la soluzione di gran parte dei problemi. Infatti, grazie al lavoro svolto dalle Autorità di bacino e dalle Regioni nell'ambito della predisposizione dei piani per l'assetto idrogeologico che prevedono la mappatura delle zone con diverso grado di rischio e pericolosità (frana, alluvione, valanga), è ormai stato delineato anche il quadro degli interventi e delle necessità finanziarie per la sistemazione idrogeologica del territorio nazionale. Tale quadro mostra che il Paese è chiamato ad affrontare, nel breve periodo, un impegno economico di oltre 10 miliardi di euro, a cui si aggiunge un impegno di oltre 30 miliardi di euro nel medio e lungo periodo.

per cento dei Comuni italiani). Per coniugare l'esigenza di sviluppo economico e sociale con quella di garantire la sicurezza degli abitati e delle infrastrutture è necessario, in primo luogo, procedere alla realizzazione degli interventi previsti nei predetti piani. Al riguardo, si fa presente che i fondi per la difesa del suolo erogati dai Ministero dei lavori pubblici tra il 1991 e il 2003 e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra il 1998 e il 2007 sono stati di circa 5,6 miliardi di euro, dei quali circa 2,5 miliardi, relativi al periodo tra 1998 e il 2008, per interventi urgenti. A questi si aggiungono i fondi per le aree depresse e quelli degli accordi di programma quadro per la difesa del suolo per circa 1,5 miliardi di euro, relativi al periodo tra il 1998 e il 2008, ripartiti secondo le necessità strategiche di sviluppo regionali. Complessivamente, dal 1991 al 2008, lo Stato ha investito circa 7 miliardi di euro per il finanziamento di interventi di difesa del suolo. Purtroppo, questa dinamica di sostegno alla spesa per la difesa del suolo, per quanto significativa, appare piuttosto modesta a fronte delle esigenze idrogeologico e considerate necessarie per portare il Paese fuori dall'emergenza da rischio idrogeologico. Inoltre, è necessario affinare la capacità di previsione degli eventi ma, naturalmente, non ci si può limitare alla gestione dell'emergenza. La prevenzione delle calamità comporta la necessità di realizzare interventi strategici. La pianificazione va connessa a misure volte a compensare i vincoli ed a sollecitare la partecipazione di capitali privati, nonché ad incentivare la delocalizzazione di manufatti, le iniziative in campo agricolo e gli interventi di riforestazione compensativa nei bacini idrografici, in modo da riequilibrare i finanziamenti verso la prevenzione e l'intervento ordinario.

ma si tratta di piccole comunità molto laboriose, che non sono in grado di provvedere per proprio conto al reperimento delle risorse finanziarie necessarie a far fronte a danni che, collocati in tale contesto,

Oltretutto bisogna tener presente che queste zone sono state duramente colpite prima di Natale proprio da un terremoto violento, tant'è vero che questo Governo ha riconosciuto i danni subiti in particolare dalle strutture religiose e storiche di quella zona,

milioni di euro. Con questo voglio dire che siamo consapevoli che questa particolare zona del parmense non è nuova a frane e smottamenti dovuti alla piena del fiume; di certo gli abitanti di queste località ricorderanno anche l'inondazione che anni fa ha causato anche la morte di alcune persone. Il rischio idrogeologico è chiaramente condizionato in maniera forte dall'azione dell'uomo e dalle modifiche del territorio. La Provincia di Parma è stata oggetto nell'ultimo decennio di diversi studi specialistici,

straripamento del 7 giugno, è costituito dal ponte Roboni. Il ponte, attraversato dalla provinciale nelle vicinanze delle località oggetto dello straripamento del fiume, è stato costruito con una portata inferiore rispetto a quello situato a monte. Ciò crea un inevitabile effetto imbuto che è causa

Comunico che sono pervenute alla Presidenza mozioni e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Grazie